Comunico che in data 11 novembre 2016 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*: «Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»

chi non rispetta una sentenza di un giudice è sicuramente soggetto a gravi sanzioni, quantomeno all'esecuzione forzata di quanto stabilito dal giudice. Quale giudice più alto della Corte costituzionale? Paese la Corte costituzionale, con una sua sentenza, ha stabilito a suo tempo che era incostituzionale la norma approvata nel 2011

forse anche meno - di quanto la Corte costituzionale ha stabilito. Come definiamo uno che non applica le sentenze di un giudice? Tutto tranne

Contro questo decreto-legge sono stati presentati vari ricorsi da parte di persone che sono state colpite da tale provvedimento e che non hanno ricevuto quanto la Corte costituzionale aveva stabilito. Mi sembra abbastanza probabile che la Corte costituzionale intervenga, però non si sa, perché la Corte costituzionale nel frattempo ha un po' cambiato fisionomia, per cui potrebbe anche assumere delle decisioni un po' diverse. tanti pensionati che si aspettano giustizia, ed è vero che la giustizia l'hanno già avuta, perché la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla base di ricorsi che sono sicuramente costati tempo, fatica e denaro: denaro: evidentemente, preparare i ricorsi e portarli avanti nelle varie istanze fin davanti alla Corte costituzionale ha i suoi costi; ma di fronte a questi costi il Governo è inadempiente.

applicare pienamente la sentenza n. 70 del 2015, la quale stabilisce che gli adeguamenti al costo della vita devono essere corrisposti nella misura che ha stabilito la Corte costituzionale e non in quella che, "a capocchia", ha deciso il Governo.

i mutui e i prestiti di cui si devono far carico gli aspiranti pensionati. Questi ultimi non è che vogliano andare in pensione giusto perché hanno fretta di andare a pescare anziché andare al lavoro, ma perché magari hanno perso il lavoro e non sono in grado di trovarne un altro, anche per questioni di età. Inoltre, chiediamo un aumento delle pensioni per i soggetti disagiati e di ridurre il livello di tassazione dei trattamenti pensionistici. Ridurli in che modo? Tanto per cominciare, ce ne sarebbe uno molto semplice, che sarebbe anch'esso un rimedio a una palese incostituzionalità di un altro provvedimento, e cioè e cioè cessare la discriminazione per cui, tra due persone a parità di reddito, il dipendente - naturalmente se ha determinati requisiti - prende i famosi 80 euro, mentre il pensionato no, e questo è palesemente incostituzionale. Solo che anche in questo caso non si è riusciti ancora ad andare davanti alla Corte costituzionale con un ricorso in proposito, anche perché i costi sono certi ma i benefici incerti, visto che il Governo non applica le sentenze C'è un'altra cosa che non dipende da noi: l'esito del *referendum*. Mi sembra chiaro che un pensionato che voglia mettere una croce sugli arretrati che gli spettano ha una via molto breve per farlo: votare sì al *referendum*, così avremo

Con una Corte costituzionale al servizio del Governo queste cose possono succedere. Invece, se non passa il *referendum* avremo ancora una Corte costituzionale indipendente, con tutti i suoi limiti, naturalmente, ma indipendente. Credo che questa sia una tutela per tutti: oggi è una tutela per i pensionati, domani potrà essere una tutela per chiunque altro. In altre parole, avere istituzioni sane che funzionano bene serve anche nelle questioni molto pratiche come, ad esempio, ricevere quanto spetta di pensione (e quanto spetta non secondo i calcoli del pensionato, ma secondo quanto ha stabilito nientemeno che la Corte costituzionale). Vorrei vedere se altri Governi avessero violato in modo così aperto una sentenza della Corte costituzionale cosa sarebbe successo: un putiferio, «l'illegalità», «la democrazia calpestata», «i giudici della Corte costituzionale calpestati». L'ha fatto il Governo Renzi e, a quanto pare, questo non crea grossi problemi alla grande stampa, che sostiene il Governo; non crea grossi problemi alle forze politiche di Governo; crea però un grosso problema ai pensionati che si vedono derubare del frutto del loro lavoro.

illustro anche io una proposta di mozione che muove dalle considerazioni che il senatore Malan ha appena svolto. Dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quel provvedimento sulla perequazione

ne sono stati esclusi dalla rivalutazione ben 5.242.161: vale a dire un pensionato su tre. Successivamente alla sentenza, il Governo è intervenuto con un decreto-legge, procedendo ad una parziale, parzialissima - pari a circa il 10 per cento - restituzione degli a una limitata ricostruzione dei trattamenti pensionistici. Ciò non era proprio corretto perché, in conseguenza di ciò, migliaia di cittadini, vedendo violati i loro diritti

perché oltre alla sentenza della Corte i tribunali di Brescia, Milano, Palermo e Genova, la Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, delle Marche e dell'Abruzzo hanno accolto i ricorsi dei cittadini contro l'INPS, facendo espresso riferimento alla giurisprudenza costituzionale.

non si discosterà da quanto affermato nella precedente sentenza n. 70, avendo già allora rilevato come siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto e del trattamento stesso e irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. In questa sentenza c'è di qualsiasi politica riferita alle pensioni che possiamo considerare equa, giusta, proporzionale e ragionevole. Dunque, la nostra proposta di mozione chiede in primo luogo la piena attuazione della sentenza della Corte, ovvero che sia rispettato il diritto acquisito dai cittadini in materia di pensioni. Per questo chiediamo di darne piena attuazione, oltre che per essere fedeli e leali al principio che una sentenza della Corte costituzionale non può che essere immediatamente applicata.

una questione di scelte. È chiaro che il tema delle pensioni richiede un approccio strutturale e di ampia visione, capace da un lato di garantire la sostenibilità, ma, dall'altro, anche la dignità dell'uscita dal lavoro. Dico questo, signora Presidente, sapendo di avere in lei un'attenta ascoltatrice su temi come questi, soprattutto pensando alla debolezza strutturale della contribuzione femminile, che trascina sul fronte pensionistico tutte le difficoltà che già incontra nel mercato del lavoro. Il punto però per tutti è quello dell'adeguamento strutturale della pensione minima al costo reale della vita. Al riguardo va ricordato come l'aumento dei trattamenti, introdotto dal Governo Berlusconi il 1° gennaio 2002, portò l'assegno dai precedenti 392 euro a 516 euro al mese. È doveroso chiedersi oggi se, alla fine, al cittadino che percepisce una pensione minima convenga di più percepire la quattordicesima, come leggiamo nei più recenti interventi del Governo, o vedersi aumentato il trattamento minimo, che nel corso di questi quattordici anni - ben quattordici anni - non è stato adeguato. Noi riteniamo sia meglio che il cittadino debba vedere adeguata la pensione al reale costo della vita, perché la somma mensile che andrebbe a percepire rappresenterebbe sicuramente su base annuale un aumento ben più elevato elevato di quello che il Governo si prefigge di erogare con la sola quattordicesima. Non vorrei, quindi, che questa quattordicesima, che suona così bene, alla fine dei conti mozione chiediamo di riformare il sistema pensionistico secondo le caratteristiche del mercato del lavoro, mettendo in sinergia le politiche a favore dell'occupazione, delle imprese e delle famiglie, e delle famiglie, prevedendo, come primo pilastro, l'istituzione di un trattamento di base, uguale per tutti e ragguagliato all'importo dell'assegno sociale da adeguarsi con cadenza periodica al costo della vita, un secondo pilastro, con versamenti effettuati sulla base di un'aliquota contributiva uniforme pari al 25-26 per dipendenti e autonomi, che diano luogo ad una pensione obbligatoria di natura contributiva, come terzo pilastro, il finanziamento di un'eventuale pensione complementare, dove il lavoratore possa optare per il versamento volontario della corrispondente quota contributiva di alcuni punti non versata alla previdenza previdenza obbligatoria INPS. perché sono certa che, trattandosi di un tema che trasversalmente interessa tutti, *in primis* un Governo che vuole indicare ai propri cittadini una strada futura positiva, non possa che accogliere le mozioni presentate stamane dall'opposizione.

non è organizzato in forma contributiva: il sistema contributivo è stato introdotto solo per la quantificazione di alcuni trattamenti previdenziali. il sistema pensionistico italiano interviene a soddisfare un principio contenuto nella nostra Costituzione, in modo particolare nell'articolo 3, quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Tale dettato è accompagnato dal principio, sempre contenuto nella nostra Costituzione, di garantire a tutti i cittadini una vita libera e dignitosa. Su questo principio si fonda anche il trattamento previdenziale cosiddetto minimo, cioè quello destinato ad assicurare la sopravvivenza ma, come ho detto, la nostra Costituzione impone

emesse dalla Corte costituzionale in materia di adeguamento dei trattamenti previdenziali, ma soprattutto richiamarlo a corrispondere a questo principio, partendo dal presupposto che gran parte delle condizioni di povertà sono connesse proprio ai trattamenti previdenziali e ai trattamenti previdenziali minimi. Nel 2015 si considerano 1.582.000 le famiglie in condizione di povertà assoluta:

di povertà assoluta. Quante di queste vivono la loro condizione anche dopo anni di lavoro di lavoro scarsamente retribuito, spesso vissuto in modo precario e che non ha dato la possibilità di maturare una previdenza del lavoro certa

previsto un aumento delle pensioni minime, portando il valore dell'assegno mensile al di sopra della soglia di povertà, quindi all'incirca a 1.000 euro netti, intervenendo in questo anche con una riduzione del prelievo fiscale (si è parlato,

come un appello al Governo: le organizzazioni sindacali, il sistema associativo, dove si organizzano gli interessi più vivi delle persone, vanno recuperati. Abbiamo bisogno di interloquire

della crisi, il tentativo di uscirne e di ridurre il debito pubblico del nostro Paese. Penso che quella sia stata una strada sbagliata, che ha determinato una contrazione della spesa pubblica per consumi che ha causato, a sua volta, una contrazione della capacità produttiva del Paese e penso che su quella strada si debba ritornare per rivedere la legge Fornero e i suoi effetti tutti (per citarne uno, quello relativo alla cosiddetta "quota 96" dei lavoratori della scuola), anche per consentire a questo Paese di procedere verso una modernizzazione attraverso l'immissione nel mercato del lavoro di tanti "giovani". Parlo di giovani tra virgolette, perché sono soggetti ormai

tra coloro che vivono una condizione di lavoro precario - i giovani - e incontrano grandi difficoltà nell'ingresso del mercato del lavoro pur avendo qualità sicuramente importanti e coloro che provengono da un mercato del lavoro che è stato progressivamente impoverito sotto il profilo delle garanzie e quindi delle speranze e degli stimoli a fare meglio, a fare di più per dove si lavora, per chi si lavora, per come si produce e per chi si produce, ma anche per l'intero Paese.

fondata sul lavoro» perché individua proprio in questa categoria di soggetti sociali, coloro che si dedicano alla produzione della ricchezza, la vera ossatura e la spina dorsale del Paese e anche le speranze di crescita del nostro popolo.

Signora Presidente, gentili colleghi, dal presidente Renzi sono arrivati annunci di importanti revisioni del sistema pensionistico, a cominciare da dove ve n'è più bisogno, ovvero nella platea dei milioni di anziani costretti a vivere con poco più di 500 euro al mese. Vorrei che per un attimo tutti voi vi soffermaste a pensare cosa significa condurre un'esistenza con 500 euro al mese, magari dopo una vita di fatiche. 500 euro al mese vuol dire vivere con 100 euro a settimana, con cui a volte bisogna acquistare medicine, oltre che pagare le bollette.

Ricordatevi che un giorno sarete vecchi anche voi e magari qualcuno si arrogherà il diritto di farvi vivere con 500 euro al mese. Voi sareste in grado? Sarebbe ingiusto? E perché invece è giusto per quei milioni di italiani e italiane che devono fare i conti tutti i giorni Purtroppo, al momento non sappiamo ancora quale sarà l'effettivo impatto della riforma delle pensioni, dato che la manovra è all'esame e al vaglio del Parlamento e la Commissione europea chiede anche modifiche al ribasso rispetto a quanto contenuto

Il problema innegabile è costituito dalla riforma Fornero, che ha prodotto un devastante sciacallaggio: oltre che andare in pensione sempre più tardi, i pensionati hanno anche perso buona parte del loro potere d'acquisto, diventando sempre più poveri. Sappiamo bene che più si invecchia, più si ha bisogno di cure e assistenza, che tanti dei nostri anziani non si possono più permettere. Sono inorridita, quando una deputata collega ha detto che, se hanno bisogno, i nostri anziani si possono ipotecare la casa.

Per non parlare poi, delle persone rimaste intrappolate in un sistema lavorativo distorto, le quali si sono ritrovate sfruttate dai loro datori di lavoro senza che questi ultimi abbiano pagato loro i contributi, e che ora, a sessant'anni, si ritrovano con un pugno di mosche in mano. E poi, non nascondiamolo: è a dir poco ridicolo doversi indebitare a sessantatré anni per pagare i contributi per la pensione, dopo anni di fatiche e sacrifici passati a lavorare. Se proprio vogliamo restare con i piedi saldi a terra e guardare in faccia la realtà, non dobbiamo dimenticare che, oggi più che mai, con l'imperversare della crisi, le pensioni dei nonni sono il principale ammortizzatore sociale delle famiglie colpite dal dramma della disoccupazione, sopratutto quella giovanile. Ancora una volta, chiediamo al Governo di intervenire con forza e operare tagli alle pensioni così dette d'oro e per aiutare chi vive con le pensioni minime. Con la mozione che il Movimento Fare! ha presentato impegniamo il Governo a reperire le occorrenti risorse finanziare per riconoscere, sia pure con un criterio di gradualità nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo in favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco l'integrale e totale restituzione ad intervenire sulle cosiddette pensioni minime non soltanto in termini di riduzione della tassazione, ma anche in termini di aumento dell'importo del trattamento, al fine di consentire un effettivo recupero del potere di acquisto dei percipienti l'assegno previdenziale, in relazione all'andamento reale del costo della vita. poi di adottare gli opportuni provvedimenti normativi affinché ai titolari di pensioni minime sia riconosciuta una maggiorazione di importo in proporzione ai contributi silenti, comunque versati nell'arco della vita lavorativa e non conteggiati sul trattamento, di ripristinare la corretta gerarchia sugli istituti di patronato, legittimati ad operare, in base alla legge n. 152 del 30 marzo 2001, a tutela degli interessi della parte debole, cioè i pensionati, sotto le direttive del Ministero del lavoro. Per questo, gentili colleghi, vi invito ad uscire dalle retoriche della propaganda pseudo-elettorale e chiedo al Governo di accogliere la mozione del Movimento Fare! che non fa altro che chiedere quell'equità di cui tutti si riempiono la bocca.

la questione pensionistica è finalmente al centro del dibattito politico. Poc'anzi ho ascoltato l'intervento del senatore Uras, di cui ho grande stima e rispetto, per la serietà che mostra verso le idee di cui è portatore, e devo contestare alla radice quello che il senatore ha poc'anzi detto, ovvero che, sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, il sistema pensionistico italiano basato sul sistema contributivo, ovverosia che le pensioni di questa Nazione dovrebbero essere elementi figurativi e non agganciati alla contribuzione del singolo cittadino.

nei termini in cui l'ha letto e interpretato il senatore Uras, creerebbe cittadini di serie A e cittadini di serie B. Infatti, i milioni di lavoratori autonomi in questa Nazione hanno tutti, senza eccezione alcuna, una pensione che è esattamente lo specchio del contributo che durante l'attività lavorativa hanno versato. ci sarebbe un articolo 3 dedicato ai dipendenti statali o ai dipendenti della pubblica amministrazione, che non vale, come tutela generale, per i lavoratori autonomi. Vorrei, invece, dire al senatore Uras che la riforma della Costituzione è necessaria non tanto per il bicameralismo, ma perché questa Costituzione, frutto di un compromesso tra le forze socialcomuniste e quelle cattoliche e liberali, ha nei suoi articolati, in funzione del compromesso, norme che si possono leggere e interpretare in maniera diametralmente opposta. Per me, l'articolo 3 significa l'uguaglianza delle opportunità, non l'uguaglianza di essere assistiti attraverso istituti pensionistici.

Né l'articolo 1 - che è un'altra grande scemenza, frutto di quel compromesso - può essere inteso come lo interpreta il senatore Uras, perché il lavoro non appartiene ai principi generali: è come dire che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla buona salute dei cittadini. I valori grandi, i valori supremi sono il progresso e la libertà, non la salute o il lavoro. Questo per dire che che quella lettura dell'articolo 3, quella demagogia socialcomunista, ha portato il sistema pensionistico italiano a riconoscere a 7 milioni di pensionati statali retribuzioni che vanno oltre i contributi versati.

questo vale 93 miliardi di euro l'anno. Questi 93 miliardi - non i 130-140 milioni della propaganda becera contro gli stipendi dei parlamentari - che lo Stato si permette di erogare

ebbene, qualche giorno fa, il presidente dell'INPS ha detto che, così come stanno i conti, le future generazioni dovranno lavorare fino a 75 anni per poter percepire una pensione, perché, se dal salvadanaio c'è chi prende il 60 per cento in più di ciò che mette, significa che i nonni e i padri stanno rubando e mangiando la pensione ai nipoti. Si possono dire queste verità lapalissiane? Possiamo dire che in questa nazione c'è un milione e mezzo di *baby* pensionati che ci costano 10 miliardi Possiamo dirle, tutte queste cose, o dobbiamo sempre fingere di non sapere, lamentandoci ipocritamente dei 480 euro che diamo ad un pensionato? Se non c'è perequazione, se c'è ancora quest'idea che lo Stato debba avere una funzione sociale e assistenziale, così come ce l'ha descritta il buon Uras, l'istituto delle pensioni in questa nazione funzionerà nel modo seguente: i lavoratori autonomi sono i fessi della situazione e prendono esattamente quello che mettono nel salvadanaio, salvo che il Governo non metta le mani anche sulle casse di previdenza; i lavoratori pubblici, in questo momento, sono quei 7 milioni che fino ad un certo momento prendono la pensione calcolata sull'ultimo stipendio e che ci costano circa 93 miliardi in più; poi ci sono i lavoratori pubblici che quell'istituto non lo vedono più applicato (come nel nostro caso, dove non ci sono più vitalizi, ma pensioni contributive) e che quindi hanno perso quel privilegio;

Chi è che non vuole dare di più ai bisognosi? Ma poiché non c'è alcun pranzo che non sia pagato da qualcun altro, quando fate i filantropi ci dovete dire dalle tasche di chi volete prendere i soldi perché, se sono sempre gli stessi a pagare, i filantropi sono i contribuenti che cacciano i soldi, non il senatore Uras, che invoca una funzione salvifica dello Stato assistenziale e clientelare

Per quanto ci riguarda, va applicata la sentenza n. 70 del 2015, perché se abbiamo tolto a quelli che percepiscono pensioni pensioni oltre sei volte il minimo, probabilmente abbiamo fatto bene, ma la Corte costituzionale dice che ci sono dei diritti acquisiti.

e noi non ci troviamo più in queste condizioni, ma non deve essere la Corte a stabilire in punto di diritto che il diritto è flessibile a seconda del risparmio che il Governo intende recuperare: se c'è da restituire quello che è stato malamente tolto, va restituito a tutti quanti, anche a quelli che prendono più di sei volte. Anche perché questa piramide va assottigliandosi mano a mano che andiamo in alto e, quindi, il risparmio complessivo è scarso. Ma in questa nazione deve valere il diritto, non il calcolo del Ministro dell'economia Pertanto, la nostra mozione si fonda su questo criterio: che a tutti sia restituito il maltolto e che vengano adeguate le pensioni minime, anche non riconoscendo più un diritto, come è stato fatto in questo caso, a quella parte di persone gratificate nel tempo delle vacche grasse da uno Stato Pantalone, per destinare quelle risorse agli ultimi e ai bisognosi. Questa è la vera giustizia distributiva, non altro.

di esame del decreto-legge n. 65 del 2015, a seguito della famosa sentenza n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione». Questa è una parte della sentenza n. 70. nel richiamare il legislatore al rispetto dei parametri costituzionali di proporzionalità e adeguatezza in materia di diritti connessi al rapporto previdenziale, fa presente che non è stato ascoltato il monito della sentenza n. 316 del 2010 su due questioni principali: *in primis*, il fatto «che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure

genericità della disposizione censurata nell'indicare quali fossero precisamente le esigenze finanziarie, per le quali il legislatore indicasse un necessario bilanciamento con i diritti dei pensionati alla perequazione; tuttavia, la Corte ha più volte ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidono sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati limiti di ragionevolezza e proporzionalità: in questa ottica, infatti, la sentenza n. 70 del 2015 ha inteso rimarcare le differenze esistenti tra quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 e altre analoghe disposizioni in materia, in particolare richiamando l'articolo comma 19, della legge n. 247 del 2007, ai sensi del quale, per l'anno 2008, la rivalutazione automatica non è stata concessa ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS; si ricorda che già in precedenza erano stati introdotti meccanismi di blocco della perequazione automatica, ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale: in particolare, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 stabilì che non spettasse la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 256 del 2001 aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale disposizione, precisando che "la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, incontra il limite delle risorse disponibili. A tale limite il Governo e il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa, con particolare rigore a presidio degli equilibri del sistema previdenziale";

la sentenza n. 10 del 2015, di soli tre mesi precedente alla sentenza n. 70 del 2015, relativa alla limitazione della retroattività della pronuncia sulla illegittimità della Robin tax, ha dichiarato la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza

aver tenuto sufficientemente conto dell'articolo 81 della Costituzione e del fatto che dopo la legge costituzionale n. 1 del 2012 occorra "gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale", come affermato dalla Corte con la sentenza n. 260 del 1990; il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni va valutato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, secondo i quali,

è intervenuto sul blocco dell'indicizzazione negli anni 2012 e 2013, in risposta a una drammatica contingente situazione finanziaria, stabilendo un diverso meccanismo di indicizzazione, che ha tenuto conto delle compatibilità finanziarie al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

- discussione che abbiamo già svolto in quest'Aula - che il ripristino, *sic et simpliciter*, del precedente meccanismo avrebbe determinato oneri per 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 e per oltre 4 miliardi di euro a regime, a decorrere dal 2016, cifre incompatibili con lo stato finanziario ed economico del Paese, con il rischio di un'apertura di una procedura di infrazione per violazione delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, nonché di un grave danno per le fasce più deboli della popolazione, a cominciare dai pensionati con assegni più bassi. Di qui la scelta della politica, in base alle sentenze della Corte costituzionale. Con il suddetto decreto-legge, il legislatore ha compiuto scelte che hanno favorito, con la restituzione della mancata perequazione, i redditi medio-bassi, ovvero una platea di circa 3,7 milioni di pensionati, prevedendo - è bene ricordarlo - l'indicizzazione nella misura del 100 per cento per le pensioni fino a tre volte il minimo, nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo, nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, e non riconoscendo alcuna perequazione per i trattamenti di importo complessivo superiore a sei volte il minimo INPS.

Con la mozione in esame chiediamo al Governo di introdurre un sistema di perequazione basato sugli "scaglioni di importo", confermando, a decorrere dal 2019, il ritorno al meccanismo già previsto dalla legge n. 388

legge n. 388 del 2000; 2) a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati, volto a proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale degli stessi e a valutare la possibilità, tenendo conto dei vincoli di bilancio, di recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione *una tantum* del montante nel 2019. In sostanza la nostra richiesta si basa sulla necessità di riconoscere il diritto dei pensionati ad avere la perequazione pensionistica, ma con gradualità e proporzionalità e, soprattutto, tenendo conto dell'attuale scenario generale, in cui anche le organizzazioni sindacali

In questi anni poco o nulla si è fatto per garantire questi diritti ai cittadini italiani.

ha dichiarato illegittima la norma che escludeva per gli anni 2012 e 2013 la perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo La Corte costituzionale nella sentenza che dichiarava illegittima tale disposizione indicava come la norma oggetto della sentenza fosse lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita e l'adeguatezza

soglia. Si sbandierano così le esigenze di bilancio per non dare atto alla sentenza.

senatrice Parente, che citava nel suo intervento la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 316 del novembre 2010.

Quindi, il decreto-legge non fa lo stesso.

ancora di più se pensionato e dopo una vita di sacrifici e di lavoro. Probabilmente ha diritto a vivere tranquillamente e a potersi occupare della famiglia. Anche questo è un valore accresciuto e accresce il valore dell'Italia perché, se ci si può occupare della famiglia, si hanno famiglie più sane, si hanno nipoti che crescono in in modo più tranquillo e generazioni che possono pensare al futuro. Noi abbiamo generazioni disperate e nonni che devono risparmiare sulla propria pensione di 500 euro al mese per poter aiutare figli e nipoti che dovrebbero avere un lavoro grazie al tanto

act*, ma esso ha aumentato il tasso di occupazione solo nelle percentuali e non nei fatti reali. Ciò emerge dai dati dei consumi, che sono bassissimi e non sono aumentati. È chiaro che questo dato di leggero aumento dell'occupazione è fittizio: sono più i lavoratori che lavorano con i *voucher* che i lavoratori occupati con una vera retribuzione e con un salario dignitoso. Quindi noi chiediamo, così come abbiamo chiesto da venti mesi in quest'Aula e in Commissione lavoro (dove il provvedimento

in più il pensionato ha anche diritto al contributo per l'abitazione in caso sia al di sotto della soglia di rischio di povertà. Inoltre, voglio ricordare a quest'Assemblea che nel 2014 tra le sette violazioni della Carta sociale europea addebitate all'Italia dal Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa era stato segnalato proprio l'ammontare delle pensioni minime, che quest'Aula e questo Governo non vogliono affrontare, perché è meglio tenere sotto ricatto le famiglie italiane piuttosto

chi ha contribuito e lavorato per quarantun anni di andare in pensione lasciando finalmente il posto a quei giovani che non si meritano,

dai il posto a chi invece è giovane, ha studiato e così magari non è più costretto ad andarsene fuori dall'Italia. Infatti sono

questo vuol dire iniziare a pensare a un sistema e a un tipo di Italia davvero diverso, che pensi davvero ai propri cittadini, così come fanno gli altri Paesi europei, come ho potuto vedere con i miei occhi la scorsa settimana in Finlandia. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Assisi, in provincia di Perugia. Benvenute e benvenuti al Senato.

in parallelo anche al fatto che si cerca di voler perequare tutte le pensioni al di sopra di cifre veramente importanti, perché sopra quattro volte o tre volte il minimo non è poco. Pensiamo che oggi i dipendenti e chi ha un lavoro minimo, un operaio, guadagnano 1.300 euro, quindi molto meno di quattro volte le pensioni; se ci campa l'operaio, ci può campare in questo momento difficile il pensionato che prende quattro volte il minimo. Credo allora che effettivamente la scelta fatta nella mozione e dal Governo nel 2015, quando si decise di fare una perequazione solamente su alcuni tipi di pensione e di rivalutare solo quelle, sia la scelta più congrua.

Sono d'accordo con l'aumento delle pensioni minime, ma vanno aumentate in un meccanismo tale da dare a chi effettivamente ha necessità e non da dare spalmando orizzontalmente

Torno sempre al punto iniziale; oggi ci sono persone che lavorano e prendono sicuramente meno di tre volte la pensione minima. Mi vengono in mente tutti i dipendenti pubblici, che sono un numero molto più esiguo dei pensionati. Questi ultimi sono infatti 16 milioni in Italia e votano probabilmente per Camera e Senato, se la riforma